come tutti sappiamo, domani è la Giornata internazionale della donna. Questa data e quella del 1° maggio sono le uniche commemorate quasi universalmente, quindi è una data storica. E a questo proposito desidero ricordare che nel 1910 la polacca Rosa Luxemburg e la tedesca Clara Zetkin convocarono la celebrazione del giorno 8 marzo. Questo accadde durante lo svolgimento della seconda Conferenza delle donne dell'Internazionale socialista tenutasi a Copenhagen. La proclamarono in un caseggiato nel quartiere operaio di Noerrebro. E da qui la mia tristezza: infatti, quell'edificio avrebbe dovuto essere conservato come luogo storico fondativo dell'Europa democratica, ma così non è stato. Pochi giorni fa, dopo un brutale intervento poliziesco contro giovani e meno giovani che lo difendevano, l'edificio è stato occupato e in breve demolito sull'altare della speculazione immobiliare. Molto si potrebbe dire sulla trasformazione delle celebrazioni in icone fredde e svuotate del loro contenuto reale. Non lo faccio perché non è questo il momento. Vorrei solo ricordare il vecchio detto dalle origini del movimento operaio: che l'8 marzo è un giorno di lutto per le donne che muoiono o soffrono nelle guerre, nello sfruttamento del lavoro clandestino, sotto la pressione patriarcale. E' un giorno di festa per le grandi conquiste realizzate, e soprattutto è un giorno di lotta per il lungo percorso che ancora è necessario compiere per la conquista della felicità possibile per tutti. *(Applausi dal

Signor Presidente, colleghi senatori, dopo la riconfermata fiducia, torniamo oggi con serena puntualità ad affrontare tematiche nodali per la vita del Paese. Prima fra tutte la drammatica questione «violenza stadi», mai dimenticata e resa prioritaria per il susseguirsi dei recenti gravi episodi. La violenza, il vandalismo, gli scenari da guerriglia urbana, le scritte infamanti contro i tutori dell'ordine vanno lette anche come spia di malessere sociale, oggetto di intervento immediato. È chiaro che gli ultimi episodi di Catania e Reggio Calabria, o i ritrovamenti di Castellammare non possono più essere tollerati da un'istituzione accorta che ha il precipuo compito di prevenire il fenomeno e migliorare le condizioni sociali, di sicurezza e di ordine pubblico. Ecco la necessità e l'urgenza di convertire il decreto-legge, imposto dopo la folle notte del *derby* siciliano, ed in continuità con le riflessioni serie e profonde sancite dalle misure dettate da Pisanu. Il testo apporta delle modifiche essenziali e soprattutto mirate, intervenendo su deroghe normative in tema di sicurezza degli impianti sportivi e contemporaneamente inasprendo la disciplina dei divieti di accesso. Bene addossare maggiori responsabilità alle società sportive, limitate nel concedere facilitazioni di qualsiasi tipo ai soggetti colpiti da condanne per reati connessi. Bene prevedere circostanze aggravanti per crimini di minaccia, resistenza e violenza ad un pubblico ufficiale. Dunque, un contenuto di norme opportunamente concentrato solo su chi è soggetto attivo di violenza e che prescinde da qualsiasi valutazione sull'addestramento, sulla capacità tecnica o sulla retribuzione delle nostre benemerite forze dell'ordine. Parallelamente, voglio prendere le distanze da chi, con voce stonata e priva di sensibilità, marcia sempre controcorrente rispetto agli indirizzi generali del Governo, anche in questi casi in cui l'appartenenza politica cede il passo alle priorità sociali. Riformiamolo sul serio questo calcio: e non solo! Restituiamo il giusto valore alla cultura sportiva, che non sia più sfogo di rabbia ed insoddisfazione, bensì momento di sana competizione agonistica tra le squadre. Deve tornare

per la coralità che ha ispirato il provvedimento e lo spirito di collaborazione che ha fatto superare anche in Commissione passaggi in cui vi era un dissenso su questioni specifiche, ma in cui si è fatta prevalere la volontà di avere una indicazione unitaria da parte del sistema politico rispetto a questi fenomeni. tutto ciò nasce per larghissima parte sull'onda emotiva dei fatti che si sono verificati qualche settimana fa a Catania e, prima, in un paesino della Calabria, seppur profondamente diversi; quella condizione drammatica, che ha fortemente impressionato l'opinione pubblica, ed anche segnalato lo stato di disagio e di sofferenza delle forze dell'ordine, che con molta forza hanno reclamato indicazioni precise dal sistema politico, volendo sottrarsi a questa condizione insopportabile per cui ogni domenica, anzi non soltanto la domenica, una larghissima messe di uomini e mezzi viene impegnata e distolta da altre attività per garantire il normale svolgimento delle partite di calcio. Tuttavia, se la vicenda di Catania ha ulteriormente allarmato l'opinione pubblica ed evidenziato il disagio delle forze di polizia, questo non ci sorprende perché è soltanto l'anello finale di una catena di accadimenti, di vicende che anche in passato fatto emergere il grave stato di sofferenza del sistema calcistico nel nostro Paese. Infatti, il Governo precedente e il Parlamento avevano definito una normativa incisiva rilevante, che noi chiamiamo in modo semplificato «decreti Pisanu». Se vi è un torto che appartiene a tutto il sistema, da quello centrale alle autonomie locali, è l'aver ritardato colpevolmente l'applicazione puntuale di quei provvedimenti; se c'è un punto di partenza obiettivamente convincente in questo decreto‑legge,

sistema giuridico sono poi vigenti concretamente nell'ordinamento. È accaduto il fatto (che a volte il vice ministro Minniti, che oggi non è in Aula, ha evidenziato con qualche imbarazzo) che attività che le società di calcio e gli enti locali dichiaravano impossibili da realizzare, se non in tempi lunghissimi, all'interno di questa condizione di emergenza e con il timore di perdere benefici, incassi e credibilità, sono state realizzate in pochissimi giorni, e quindi con l'insegnamento virtuoso che se vi è una determinazione forte

all'interno degli stadi, e nella specificità degli stadi, con una serie di norme importanti, alcune relative all'ordinato svolgimento delle competizioni calcistiche, che cercano di evitare le condizioni nelle quali gli scontri possano svilupparsi, altre che hanno l'obiettivo di sanzionare con maggiore efficacia i comportamenti in violazione delle norme. Vi è qui qui un elemento che voglio evidenziare, non per ragioni polemiche ma perché ieri il Parlamento, in una delle votazioni più importanti, si è contraddetto.

di violenza, non soltanto nelle competizioni calcistiche, ma anche in altre vicende che spesso vedono le forze dell'ordine - a cui tutti rivolgiamo apprezzamento e stima e a cui garantiamo sostegno e strumenti per la loro attività di repressione repressione - oggetto, in molte manifestazioni, di aggressioni fisiche e verbali, la reintroduzione del reato di oltraggio in alcune circostanze potrebbe costituire un elemento di prevenzione molto forte perché impedisce inibisce l'*escalation* che può arrivare anche al confronto e al contatto fisico tra forze dell'ordine e frange di contestazione o di violenza.

non prevede una sorta di chiusura attraverso la reintroduzione del reato di oltraggio. Tuttavia, accanto all'intero architrave di questo provvedimento, che riguarda le competizioni calcistiche, il controllo degli stadi,

in altri ambiti. Dunque, un'analisi attenta e puntuale di questo malessere non può essere ritardata. Vi è stata una interessante riflessione che riguarda il futuro del calcio, il ruolo e le responsabilità delle società di calcio, il problema degli impianti, di quale deve essere la loro gestione e non soltanto il loro adeguamento strutturale per consentire condizioni di sicurezza e di fruizione, ma anche il tema inerente a una a una responsabilità piena e assoluta delle società oggi evocata attraverso il ruolo degli *steward*, quindi il controllo di sicurezza che per il futuro prefigura

qualche cautela. C'è però un'altra questione che è stata evocata nelle audizioni e che rimane come elemento più importante con cui fare i conti, ed è quella che riguarda le ragioni del disagio che frange giovanili di aree territoriali e sociali diverse esprimono attraverso questa violenza inaccettabile che spesso come riferimento passivo ha le forze di polizia di questo Paese. È un disvalore gravissimo, ma è anche qualcosa di più: è una preoccupazione che deve interrogare e impegnare non soltanto l'analisi sociologica, importante per individuare gli strumenti di intervento in termini di prevenzione,

Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi siamo chiamati a votare può essere l'occasione di voltare pagina rispetto ad uno stato del nostro calcio molto grave. Può essere l'occasione per iniziare un cambiamento profondo e speriamo che questo percorso sia compiuto con senso di responsabilità e di coesione da tutte le forze politiche, con un'unità d'intenti che oggi registriamo con soddisfazione e che speriamo possa proseguire nel tempo su questo terreno. Sarà chiaro a tutti, infatti, che quello di oggi è un importante passo ma che la repressione della violenza non si può fermare a questo primo intervento emergenziale. Dobbiamo ammettere che desta stupore come, mentre le Aule parlamentari sono impegnate in una riflessione seria sul futuro del calcio e sulle strategie per fermare la violenza, fuori di qui sembra che non sia avvenuto nulla quel 2 febbraio scorso di fronte allo stadio di Catania. Non vogliamo criminalizzare nessuno, ma quando vediamo certe scritte sui muri contro le forze dell'ordine o quando sentiamo dire che lo spettacolo deve continuare, pare evidente che una parte del mondo che gravita intorno allo sport e al calcio non ha colto la serietà del momento. Noi daremo un deciso sostegno a questo provvedimento non solo per il merito, che ci convince, ma anche per il metodo. Il lavoro di tutto l'arco costituzionale e del Governo ha consentito di apportare miglioramenti profondi a quello che era già un buon testo di partenza; penso, oltre al tema della responsabilità degli organi di comunicazione, alle norme più solide in materia di nominatività dei biglietti, all'avvio della discussione sul ruolo della scuola nella costruzione di una sana cultura sportiva. Ci sembra giusto restituire alle diverse istituzioni il ruolo che a ciascuna compete. Noi siamo e saremo rigorosi nel rispetto dell'autonomia dello sport. Riterremo qualunque commistione un errore grave, ma questo non ci solleva dalla responsabilità di definire come legislatori il confine delle regole della convivenza ed il confine dell'etica dei comportamenti socialmente accettabili. Con il provvedimento oggi al nostro esame, che spero godrà di un consenso vasto, cominciamo ad affermare che i comportamenti violenti non fanno parte della cultura dello sport e non hanno nulla a che vedere con i valori che allo sport sono legati. Ora il Governo, il potere esecutivo e tutte le istituzioni, compresa la magistratura, hanno il dovere di garantire un'applicazione rigorosa di queste norme. Quello che non potremmo accettare sarebbe assistere, magari tra qualche anno, ad altri eventi drammatici come quelli che hanno scosso il Paese in queste settimane. Il Parlamento ha fatto la propria parte, quella di definire le norme. Ora non ci sono più alibi ad una repressione forte della violenza. Ma spero che sia nella consapevolezza di tutti che quello di oggi è il primo passo anche per noi. È necessario completare questo disegno complessivo: diversi interventi, di maggioranza e opposizione, hanno richiamato il tema importante della proprietà degli stadi e il ruolo che possono svolgere i professionisti della sicurezza negli impianti durante lo svolgimento degli eventi sportivi. Resta però aperto il tema degli investimenti sull'impiantistica per portare tutte le strutture ad un livello adeguato. Nessuno di noi dimentica che il calcio non è fatto solo dalla serie A e dalla serie B, e nessuno di noi, mentre ricordiamo commossi l'ispettore Raciti, può e deve dimenticare la storia di Ermanno Licursi, il dirigente morto a Luzzi, in provincia di Cosenza, durante lo svolgimento di una partita delle serie minori. E' una riflessione che avremo modo di affrontare presto, spero fin dalla discussione sul provvedimento sui diritti TV degli eventi sportivi. Se il principio della mutualità è quello che deve definire la distribuzione delle risorse tra i vari soggetti aventi titolo, il tema della sicurezza non può essere dimenticato. Oggi ci troviamo quindi ad affrontare, con spirito responsabile, un tema che non possiamo eludere e che ha attraversato il nostro dibattito come una sorta di fiume carsico; mi riferisco alla riflessione che intende lo sport solo come un pezzo dell'economia reale o anche o soprattutto come prioritario tratto sociale e identitario della Nazione. Siamo convinti che per raggiungere l'obiettivo di battere la violenza siano necessari interventi complessi; non vorremmo che passata l'emergenza i legittimi interessi e le culture che ciascuno di noi rappresenta divengano un limite al linguaggio comune che oggi parliamo. Penso alla mutualità nella redistribuzione delle risorse legate ai diritti TV, o alla già citata proprietà degli stadi in capo alle società sportive. Ci auguriamo che questi temi verranno affrontati condividendo, come esito, la promozione della cultura sportiva e dei suoi valori, non la promozione solo della ricchezza delle società sportive. Un atteggiamento fondato sulla centralità del mercato non ha funzionato, e ha mostrato le conseguenze più nefaste proprio quella sera nello stadio di Catania. Uno sport televisivo, fondato sulla competizione fuori dalle regole, in cui sia accettata una impunità di fatto sarebbe un danno per il Paese, non una risorsa. Noi invece abbiamo l'obbligo di riaffermare i valori dello sport. Non solo per un indistinto principio etico, ma per la consapevolezza delle conseguenze delle nostre scelte: uno sport malato produce e rafforza gli elementi di disgregazione sociale e funge da catalizzatore di forme di devianza sempre più aggressive. Sta alla nostra responsabilità definire regole che non si limitino a reprimere la violenza, ma che siano in grado di restituire allo sport quella funzione di promozione sociale e di educazione collettiva che ci ha tanto appassionato e che riscopriamo nei momenti felici della vita sportiva, dalle piazze piene per festeggiare la nazionale in Germania al tifo composto e appassionato per la prima sudatissima vittoria dei nostri rugbiysti contro la Scozia. Per questo continuiamo a richiamare la necessità di un intervento di vasta portata, che coniughi repressione e promozione della cultura sportiva. Solo così onoreremo la memoria di chi ha dato la vita solo poche settimane fa. Ed è con la speranza che questo percorso sia largamente condiviso che oggi il Gruppo Insieme con l'Unione voterà a favore di questo primo, importante provvedimento, comprendendo ed essendo anche convinti che

riuscire a lavorare con la stessa abnegazione, con lo stesso spirito di sacrificio che abbiamo dimostrato. Solo tenendo insieme sia la regola che l'emozione possiamo riappropriarci anche di un'autenticità del valore e trasmettere tutto ciò ai giovani.

dal contesto in cui ci siamo mossi, sicuramente possiamo definirlo condivisibile, anche se - a nostro parere - perfettibile. Noi abbiamo tentato di proporre una serie di

ma va a disdoro soprattutto di chi nel Paese non è in grado di far applicare le leggi esistenti. Ho ricordato più volte che il Governo precedente, il Governo Berlusconi, si era occupato fin da subito della tematica

di vasti strati della cultura italiana, non arriveremo mai a risolvere il problema. Il problema è questo: che esempio diamo ai tifosi? Abbiamo visto che molto probabilmente - almeno in base a quello che sembra essere l'orientamento degli inquirenti - chi ha ucciso quel povero agente è un minorenne; quindi, un ragazzo che, sicuramente, non è preparato, né dal punto di vista culturale, né da quello psicologico, ed è facilmente influenzabile.

Nessuno dei devastatori è stato assicurato alla giustizia né è sotto processo, ma, in compenso, decine e decine di esponenti delle forze dell'ordine sono processati perché colpevoli di aver tentato di difendere la città. E poi, ancora, abbiamo visto l'esempio di Oreste Scalzone, un latitante, che è tornato nel Paese non pentito e senza aver scontato la pena a cui è stato condannato: è stato annunciato che verrà ricevuto, con tutti gli onori, addirittura alla Camera dei deputati. Abbiamo visto un terrorista essere chiamato nelle università ad insegnare il proprio pensiero ai giovani giovani ed un esponente politico - un deputato, che sostiene la maggioranza - dichiarare che la soluzione ai problemi di Catania sta nel collocare un numero sull'elmetto indossato dai poliziotti, in modo da poterli identificare nel caso commettano qualche errore o qualche azione non troppo commendevole.

la glorificazione continua dei cattivi maestri, ci porti ancora su questa strada. Ricordo, infine, che, in questi giorni, viene pubblicizzata

disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente la violenza negli o intorno agli stadi. Le ragioni di fondo del decreto - alcune molto chiaramente definite, altre da definire - erano sostanzialmente tre:

segue il lavoro svolto nella precedente legislatura in un contesto di emozione, dovuta a gravi fenomeni di violenza negli stadi,

UDC abbiamo potuto lavorare per l'obiettivo complessivo di questo decreto-legge, grazie al fatto che, da tempo, il partito si è strutturato in modo da avere, nell'amico onorevole Ciocchetti, una persona che, sul punto complessivo della politica dello sport, di repressione della violenza e di prevenzione dei facinorosi, ha dato indicazioni di fondo e sono lieto di constatare che la sostanza delle nostre posizioni è stata molto apprezzata dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia; di questo voglio dare atto ai relatori Sinisi e Di Lello e ai due presidenti Bianco e Salvi. Abbiamo potuto concorrere con gli altri Gruppi sostanzialmente per ottenere i tre obiettivi la repressione dei violenti, innanzitutto. Abbiamo infatti rinforzato, in modo particolarmente severo, le norme penali a tutela della incolumità dei tutori dell'ordine; questo è l'aspetto di maggior significato che il decreto-legge aveva e che, grazie anche alle nostre proposte, avrà ancora di più: coloro i quali attentano alla incolumità personale degli addetti alle forze dell'ordine sono passibili non soltanto di fatti processuali penali significativi (la flagranza viene allungata per consentire che si consideri flagranza anche il reato commesso nell'arco di quarantotto ore dopo lo svolgimento della gara), ma soprattutto vi siano violenze fisiche nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza e delle forze dell'ordine in generale. Si è trattato di una risposta non soltanto emblematica, dopo la drammatica morte del commissario Raciti; si è trattato di una risposta culturalmente significativa: vogliamo fare in modo che coloro i quali, durante le partite o subito dopo, prendono prendono le forze dell'ordine ad oggetto specifico della loro violenza sappiano che si tratta di una violenza penalmente perseguibile in modo ancora più grave della violenza nei confronti delle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni altrove. Questo è un aspetto di particolare significato: una repressione più forte nei confronti di coloro i quali commettono reati di lesioni personali gravi o gravissime ai danni delle forze dell'ordine. Sulla prevenzione, signor Presidente, abbiamo abbiamo cercato di lavorare fino in fondo per recidere quel legame che talvolta si realizza tra le società di calcio e le organizzazioni più facinorose; abbiamo ritenuto irrisorie alcune sanzioni a carico delle società di calcio che promuovono società di facinorosi per poterli considerare tifosi a loro sostegno, sia nelle partite in casa che fuori casa, ed abbiamo notevolmente aggravato le sanzioni a carico delle società di calcio che intrattengono rapporti pericolosi con i facinorosi,

Da questo punto di vista, siamo particolarmente lieti che sia stata adottata, con il parere favorevole del relatore espresso ieri qui in Aula al Senato e dal Governo, una disposizione della proposta che prevedeva e prevede un obiettivo di promozione molto forte a favore delle società di calcio che, invece, intrattengono rapporti con associazioni anche non facenti parte di quelle previste dal codice civile in senso stretto, che promuovono la cultura legalità e dello sport. Abbiamo, cioè, voluto operare contemporaneamente nel senso della prevenzione nei confronti dei facinorosi e nel senso della promozione della cultura sportiva, il tutto perché non abbiamo adottato la linea (che nessuno, per la verità, proponeva) di sola repressione dei violenti, ma abbiamo voluto dimostrare che tendiamo a distinguere radicalmente tra i tifosi, che vanno comunque tutelati e protetti, e i facinorosi, che vanno comunque scoraggiati e puniti. È una distinzione che troppe volte negli stadi non si riesce a fare fino in fondo, grazie anche al modo in cui alcuni striscioni odiosissimi

in particolare i *derby* delle grande città), ma sono le attività collegate al calcio in tantissimi stadi minori, non sempre oggetto di attenzione particolare da parte soprattutto dei parlamentari. In altri termini, abbiamo voluto dimostrare che con questo decreto non abbiamo avuto la pretesa di disciplinare, in modo definitivo, né la questione della tutela delle forze dell'ordine comunque al di fuori delle vicende calcistiche, né la vicenda calcistica nel suo insieme. Lo dico perché vi è stato un argomento molto importante, che abbiamo preferito rendere oggetto di delega al Governo in tempi molto rapidi: quello degli assistenti dentro gli stadi, che vanno sotto il nome di *steward*. Noi vogliamo operare in un senso profondo di novità: la tutela dell'ordine negli stadi grandi, medi e piccoli deve essere delle società sportive che concorrono ad organizzare la manifestazione; fuori degli stadi l'ordine pubblico è di competenza dello Stato. Ma per fare questa distinzione di fondo, che sarebbe una radicale innovazione nella struttura del nostro mondo calcistico, occorre disciplinare la proprietà dell'immobile destinato allo svolgimento della gara, non soltanto dell'Olimpico di Roma, dell'Olimpico di Torino o del San Paolo di Napoli, ma anche del piccolo manufatto in cui si svolgono le gare di calcio nelle serie minori. Occorre anche fare in modo che la tutela dell'ordine dentro lo stadio sia fatta da persone professionalmente attrezzate. Non si può disciplinare in modo ovvio la materia degli assistenti negli stadi come se fossero guardie giurate. Il problema è molto diverso, perché la guardia giurata ragionevolmente non deve occuparsi di coloro che vogliono attentare allo svolgimento della gara, mentre chi è per preposto alla tutela dell'ordine dentro lo stadio potrebbe avere a che fare con organizzazioni anche facinorose di tifosi. Questa differenza richiede una diversa professionalità e probabilmente un diverso regime giuridico rispetto alle normali vicende che possono riguardare altre forme di cosiddetta polizia privata. Ecco perché questo decreto‑legge non è soltanto un fatto marginale che riguarda un aspetto marginale della vita dello sport, ma è un provvedimento che prende atto del fatto molto emblematico che intorno agli stadi, in questo caso soprattutto a quelli più grandi, si svolge un'attività che tende alla contrapposizione violenta e che ha sempre meno a che fare con la cultura dello sport. Le ragioni sociologiche possono essere molto varie: ad esempio, vi è una sorta di sensazione di impunità per coloro che svolgono attività violente dentro o intorno agli stadi. Noi abbiamo voluto anche reprimere il danneggiamento alle cose, non genericamente considerate, ma quelle essenziali per lo svolgimento delle gare, perché immaginiamo che questo decreto si faccia carico delle ragioni per le quali il decreto Pisanu di qualche anno fa è rimasto, sostanzialmente, non del tutto attuato: dopo la reazione emotiva che aveva portato a quel decreto, si era creata, infatti, una sorta di sentimento di lassismo nei confronti dell'attuazione del decreto medesimo. Ci auguriamo che un analogo spirito di lassismo non si verifichi in questo caso e che l'approvazione della legge di conversione del decreto, molto diverso da quello che il Governo ha emanato, ma nelle linee di fondo che il Governo aveva indicato

repressione nei confronti della violenza commessa a danno degli agenti delle forze dell'ordine, della prevenzione nei confronti dei facinorosi, della promozione della cultura della legalità e dello sport. Se su queste tre linee trovassimo una convergenza che vada al di là delle manifestazioni sportive, potremmo dire che il nostro Paese ha fatto uno straordinario passo avanti. *(Applausi *(RC-SE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, il decreto-legge all'esame dell'Aula rappresenta un intervento importante per il contrasto ai fenomeni di violenza, oggi sempre più diffusi nell'ambito delle competizioni sportive. Esso nasce, come è noto, nel contesto dei tragici fatti di Catania che hanno visto la morte dell'ispettore Raciti, alla cui famiglia testimoniamo ancora una volta la nostra solidarietà, e che hanno dimostrato ancora una volta l'esigenza da un lato di contrastare e prevenire - anche, ma non solo, con gli strumenti normativi - la violenza, in ogni sua forma e dall'altro di restituire alle manifestazioni sportive, ed in particolare al mondo del calcio, la loro dignità e il loro valore sociale. Al di là dei fatti concreti da cui nasce il decreto-legge e delle ragioni di necessità ed urgenza che hanno motivato e legittimato, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il ricorso allo strumento del decreto-legge, il testo all'esame dell'Aula si muove su un orizzonte più ampio e tocca problemi di assoluto rilievo politico e sociale, come anche il dibattito in sede di Commissioni riunite ha avuto modo di evidenziare, giungendo infine a posizioni comuni e condivise, che hanno consentito di superare iniziali rilievi di criticità, sottolineati anche dal Gruppo parlamentare di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea. Sotto il profilo normativo, il decreto-legge integra, razionalizza e completa le misure di prevenzione e repressione già previste dal decreto-legge Pisanu, intervenendo con misure strutturali che accentuano le responsabilità in capo alle società calcistiche, colpendo peraltro il legame spesso presente tra i loro interessi e le frange violente di sostenitori. Gli aspetti più innovativi del decreto-legge rispetto alla normativa previgente concernono in particolare l'intervento sugli aspetti culturali del problema per promuovere una diversa e più sana cultura civica dello sport, che hanno sottolineato anche alcuni colleghi, ed in particolare la senatrice Maria Luisa Boccia. In questo senso, è importante rilevare un mutamento di prospettiva nell'approccio al problema della violenza, che emancipa l'orizzonte dell'intervento dalla logica della prevenzione declinata in termini meramente securitari per agire anche e soprattutto sul terreno delle misure strutturali, regolando in maniera più rigorosa gli impianti e quindi i luoghi e gli ambienti in cui avvengono le manifestazioni sportive, per garantire una più efficace prevenzione dei fenomeni di violenza, e favorendo una maggiore trasparenza e un maggiore controllo sull'attività delle società sportive e sui rapporti tra esse e le consorterie dei tifosi e degli ultras, in cui si annida spesso, purtroppo, il germe della violenza, della discriminazione, dell'antagonismo violento che si deve reprimere e combattere. In questa prospettiva, le misure introdotte dal decreto-legge assumono un assoluto rilievo, nella misura in cui chiamano anche le società sportive ad assumersi tutte le responsabilità che loro competono competono rispetto a simili fenomeni, per spezzare quei legami con le frange violente delle tifoserie che favoriscono la diffusione della violenza, coinvolgendo purtroppo persino i giovani che invece da tale clima dovrebbero essere protetti. E' anche chiamando le società sportive ad assumersi le proprie responsabilità che si contribuisce a costruire una cultura comune e uno spazio condiviso nel quale la prevenzione della violenza si avvalga di strumenti diversi dal diritto e dalla pena, per fondarsi invece sul reciproco e costante intervento delle forze sociali e sulla costruzione di un approccio culturale diverso, per forme e contenuti. E' quindi sul terreno della cultura e della società che si gioca davvero il tema della prevenzione della violenza, ed in particolare di quella legata alle manifestazioni sportive, in cui è strutturalmente presente, al di là delle degenerazioni patologiche, la componente dell'agonismo e della contrapposizione che riproduce ed amplifica la dialettica e lo scontro tra vincitori e vinti. Alla luce di queste considerazioni, è auspicabile che si superi e si separi, in maniera profonda, l'intervento legislativo nel contrasto alla violenza dal ricorso sistematico e simbolico al diritto penale, che - come è noto - reca in sé sempre e comunque una componente di violenza violenza strutturale e di violazione di diritti fondamentali della persona, che ne dovrebbe consigliare un uso minimalista, rappresentando davvero l'estrema *ratio* cui ricorrere quando le altre forme di controllo sociale si siano rivelate inefficaci rispetto agli obiettivi. In tal senso, gli emendamenti presentati in Commissione dal Gruppo parlamentare di Rifondazione Comunista miravano proprio a limitare il più possibile il ricorso a misure di dubbia legittimità costituzionale e ispirate alla logica di una «perenne emergenza», che dovrebbe invece affrontarsi sul terreno della prevenzione culturale, per evitare di rispondere alla violenza sociale con una forma di «violenza istituzionale». Penso in particolare alla flagranza differita, all'inasprimento delle pene, alle misure di prevenzione mutuate dalla legislazione antimafia, che costituiscono delle pene per il sospetto, irrogate in assenza di un delitto commesso. Non è certo con la logica del diritto penale del nemico e con la caduta delle garanzie dello Stato di diritto che si combatte la violenza, perché la democrazia e la legalità non conoscono amici, né nemici, ma soltanto innocenti e colpevoli e perché la violenza si combatte con la prevenzione culturale, l'educazione alla legalità e ai princìpi dello Stato di diritto, che non possono essere derogati in nome di nessuna emergenza, se davvero il diritto deve ribadire la sua differenza rispetto alla forza. Quindi, signor Presidente, onorevoli colleghi, pur testimoniando un forte disagio personale rispetto al punto di partenza che ha generato l'elaborazione del decreto in esame, che non è stato senz'altro quello di una società che si interroga sul fallimento dei propri modelli relazionali, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i fatti che hanno portato a questo decreto‑legge e alla nostra discussione parlamentare sono gravissimi: mai avrebbero dovuto accadere. Esprimiamo pertanto la nostra solidarietà alla famiglia, gravemente colpita dall'omicidio dell'ispettore Raciti, dell'ispettore Raciti, e anche a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine. La popolazione tutta, tutta l'Italia, ha reagito con ribrezzo a questo culmine in cui è sfociata la violenza, purtroppo da anni presente negli stadi. Siamo pertanto felici che dopo questi violentissimi scontri il Governo, la maggioranza, l'opposizione, tutto il Parlamento abbiano trovato una risposta forte e condivisa per emarginare queste violenti aggressioni. Una risposta che è stata discussa ampiamente nelle Commissioni competenti, in cui si è trovato lo spirito comune di porre in essere anche repressive, che veramente dia tranquillità a chi voglia andare allo stadio per divertirsi. Il sabato e la domenica sportivi devono tornare a essere ciò che devono essere, un incontro piacevole e veramente sportivo, per i giovani, per gli entusiasti dello sport e del calcio, per le famiglie. Un incontro disteso che dia spazio al vero spirito sportivo e tolga spazio a chi lo ha usato per porre in essere le proprie aggressioni.

Presidente, onorevole rappresentante del Governo, cari colleghi, gli articoli del decreto-legge in discussione e le disposizioni aggiunte dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia, che hanno operato con spirito di convergenza e con motivazioni esclusivamente rivolte a dare una risposta giusta, adeguata e condivisa anche dalle istituzioni audite nel corso della discussione, costituiscono un provvedimento moralmente e politicamente doveroso, dopo il tragico evento della morte dell'ispettore della Polizia di Stato Raciti a Catania. i contenuti degli emendamenti presentati in Aula a nome delle Commissioni riunite troviamo molti degli argomenti e delle proposte fatte dall'opposizione. Per questo voglio ringraziare i due relatori e anche il Presidente della Commissione. Questo non significa, cari colleghi, e mi riferisco alla polemica di ieri, che ci siano stati un gioco di sottobanco e di inciuci vari; non significa assolutamente questo; significa una sola cosa: quando ci troviamo di fronte a provvedimenti che riguardano l'interesse generale del nostro Paese, della nostra comunità - e questo provvedimento va posto nella categoria che ho enunciato - è doveroso per tutti quanti, anche per l'opposizione, dare il contributo.

affinché fosse delineato rapidamente un quadro di iniziative concrete, anche per rispondere ad un clima di diffusa preoccupazione tra la gente, cioè che la violenza negli stadi e fuori da essi rischia di diventare una normalità che riguarda non solo il mondo dello sport, ma tutta la nostra società. A differenza di quanto è avvenuto nel passato, di fronte ad analoghi provvedimenti adottati in conseguenza di fatti sportivi, questa volta abbiamo avuto tutti la sensazione che l'avvenimento sportivo non rappresentava la causa ma solo l'occasione per lo scatenamento di un'inaudita violenza contro le forze dell'ordine che avevano e hanno la sola responsabilità di essere tutori dell'ordine pubblico e della sicurezza della gente. Alcuni giornali, cari colleghi, parlando della tragica notte di Catania, hanno sostenuto che si trattava, in fondo, di una pagina già scritta e che avrebbe radici in un diffuso sentimento dei giovani: l'orgoglio di essere contro in ogni caso, l'esaltazione della bandiera calcistica per un protagonismo che non si riesce ad avere nella vita di ogni giorno ed, infine, anche l'estremismo politico. Altri osservatori sono di contraria interpretazione. Rifiutando ogni sociologismo, essi hanno interpretato i fatti di violenza come proiezione di un mero desiderio di realizzare piccoli ed innocui episodi di estremismo con il solo errore di averne esagerato la misura. A mio giudizio, le due tesi estreme non sono convincenti e credo che Governo e Parlamento, con il provvedimento in discussione in quest'Aula, intendono dare questa volta una forte risposta alla violenza nel calcio e nello stesso tempo anche scuotere gli animi e stimolare atto di assunzione di responsabilità di tutto il mondo dello sport dai dirigenti delle società ai giocatori, dalle curve dei tifosi agli organi di stampa, affinché lo sport non si tramuti in periodiche battaglie. In questa direzione, Presidente, va l'ordine del giorno che - devo ricordare - é stato approvato in cui noi del Gruppo di Alleanza Nazionale abbiamo chiesto l'adozione di un codice etico proprio per lo sport per il calcio per fare assumere le responsabilità a tutti i soggetti che comunque sono interessati. Il monito che intendiamo rivolgere al Paese attraverso questa legge parte dalla convinzione che è giunto il momento in cui le autorità costituite

La gente vuole anche che l'emozione sportiva e la passione non possano sconfinare in atti di criminalità contro i tutori dell'ordine, che le responsabilità individuali degli atti di aggressione e distruzione non debbano trovare giustificazione nell'impunità collettiva, che siano abbandonate tutte le tesi di giustificazione, purtroppo sostenute anche in questi giorni da qualche parlamentare che addirittura ha preteso e pretendeva che le norme sul calcio e sulla sicurezza negli stadi fossero concordati con la tifoseria delle curve. Siamo contrari a queste tesi, ma anche a quelle secondo cui il fenomeno teppistico sportivo deve essere collocato nel disagio sociale in cui vivono le giovani generazioni, come mi è sembrato di capire dalle parole della collega che mi ha preceduto. Siamo dalla parte della stragrande maggioranza dei giovani e meno che vivono e testimoniano una passione per il calcio con sentimenti di rispetto per tutti gli sportivi e soprattutto per le forze dell'ordine che tutelano l'ordinario svolgimento dell'avvenimento sportivo. Sicuramente, cari colleghi, da qualche forza politica nel Parlamento e fuori e nel Paese le norme che stiamo approvando saranno ritenute inutili o come strumento di repressione. Noi respingiamo questa accusa e siamo d'accordo con i relatori che la legge in discussione mira a fornire un quadro di norme che si colloca nella continuità del decreto Pisanu del 2003, con l'innesto di disposizioni più efficaci materia di sicurezza negli stadi, sanzioni relative alle prevenzioni, al controllo delle tifoseria, accentuando i vincoli della verifica delle identità personali degli spettatori, aggravando i divieti di accesso agli stadi per coloro che si sono macchiati di condotte pericolose per l'incolumità degli altri sportivi e delle forze dell'ordine. Anch'io ho condiviso le perplessità sull'opportunità di inserire misure di prevenzione personali e patrimoniali previste per le organizzazioni mafiose. Mi dispiace che il Governo non abbia aderito alla richiesta avanzata non solo da noi, ma anche dai

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, chiudo questo mio breve intervento annunciando il voto favorevole del Gruppo di AN. Ritengo che, come sempre, quando si discute di rafforzamento dell'autorità dello Stato, di come dare risposte immediate ad attacchi alla sicurezza del Paese, come combattere democraticamente, con la forza delle leggi, la violenza in ogni sua forma nella nostra società, AN non faccia mancare il suo contributo per iniziative legislative serie, equilibrate, incisive. Siamo convinti che questo chieda a noi il mondo dello sport, questo voglia la stragrande maggioranza delle persone perbene del nostro Paese. VIZZINI *(FI)*. Signor Presidente, colleghi senatori, i senatori del Gruppo di Forza Italia daranno il voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto del Governo, che mira a fronteggiare l'inaudita violenza che attraversa il nostro sport nazionale più popolare, del quale l'Italia è campione del mondo, ma del quale sta diventando campione del mondo anche di degenerazione della violenza. È un lungo viaggio attraverso il codice penale, quello compiuto dal calcio italiano in questi anni: dalle scommesse ai passaporti falsi;

di un arbitro rinchiuso negli spogliatoi da un dirigente calcistico alla corruzione, agli scontri tra le tifoserie e, infine, alla morte di un ispettore della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico per garantire il corretto svolgimento di una partita di calcio. Onorevoli colleghi, vorrei farvi presente che l'ipotesi di un poliziotto deceduto in un'operazione

il riconoscimento dell'opera giusta svolta dal ministro dell'interno del Governo Berlusconi, senatore Giuseppe Pisanu. Tuttavia, in questo Paese il quello dell'applicazione delle norme, dell'irrogazione delle sanzioni e delle moratorie. Nessun provvedimento di legge potrà mai avere efficacia se non viene correttamente applicato, se le sanzioni non vengono irrogate secondo quanto previsto dalla legge e, soprattutto, se si continua con eterne moratorie. Badate bene, ci sono voluti due anni pieni per non vedere negli stadi i cosiddetti tornelli per far entrare la gente assistere alle partite con un minimo di controllo; ci sono volute 48 ore per mettersi in regola, almeno per gli abbonati. È stato detto in discussione generale che ciò è avvenuto, peraltro, facendo la fortuna delle ditte che fabbricano i tornelli, le quali, ovviamente, hanno raddoppiato i prezzi; si è fatto in tre-quattro giorni, in una settimana, quello che non si era fatto in due anni, lasciando correre. Abbiamo appreso di tutto, durante le audizioni,

vi pregherei di non volgere stabilmente le spalle all'oratore. Vi prego di capire il termine «stabilmente», perché può capitare che ci si giri con le spalle all'oratore, ma stare minuti interi in quella posizione mi pare una cosa

Questo decreto contiene norme volte a fronteggiare la violenza, ma non basterebbe a nulla se esso non fosse collegato ad un processo di cambiamento complessivo delle regole del calcio nel nostro Paese. Noi facciamo qui misure di sicurezza, sistemi di sanzioni, misure di prevenzione e di polizia, ma dobbiamo guardare ad un futuro in cui cambi il sistema di funzionamento degli stadi, cioè la proprietà degli stadi, le funzioni di quelli che vengono chiamati *steward* (non capisco perché non troviamo un termine italiano per definire funzioni di polizia privata, come ci sono a salvaguardia degli aeroporti e delle banche nel nostro Paese) e anche le sanzioni, che non siano soltanto quelle di tipo amministrativo che ammontano a poche decina di migliaia di euro. Se vogliamo risanare il calcio italiano per riportarlo nell'alveo di quello che deve essere uno sport, ci vuole la collaborazione delle società di calcio, che, vedi caso, sono state le uniche delle audizioni che abbiamo svolto, si sono fatte sottorappresentare: abbiamo tenuto audizioni con i vertici del CONI e di tutte le istituzioni che abbiamo chiamato, ma non abbiamo avuto la fortuna di poter incontrare né il presidente né il vice presidente della Lega calcio, che sono gli interlocutori con cui bisogna per rompere il legame tra le società e le tifoserie, affinché gli elenchi dei tifosi facinorosi (a cui sono stati regalati per anni biglietti per le trasferte e finanche il *merchandising*, cioè l'uso del marchio delle società) vengano consegnati alla questura e alle forze dell'ordine per poter capire con chi si ha

Portando a Catania o a Bergamo 1.500 agenti della Polizia di Stato per garantire l'ordine pubblico in una partita di calcio? Credo che quando una città italiana, una società di calcio, un pezzo del territorio per far svolgere un evento sportivo ha necessità di 1.500 agenti, allora bisogna dire che non si può disputare quell'evento sportivo, perché la polizia sul territorio in questo Paese - e soprattutto nel Mezzogiorno - serve per emergenze che sono, credetemi, un po' più gravi di quella rappresentata dal corretto svolgimento di un campionato; salvo che poi il problema non sia che, siccome il sistema delle scommesse nel calcio, dei diritti televisivi, cioè il sistema di tutto quello che non si può fermare, è talmente più forte delle esigenze di una società civile di vivere correttamente, allora si chiudono gli occhi e si va avanti. Credo che nessuno di noi può volere cose di questo genere. E allora bisognerà lavorare con la Federazione italiana giuoco calcio con la Lega calcio, perché le vere sanzioni che porteranno le società a far rispettare l'ordine, esse stesse, non sono i 20.000 o i 30.000 euro di sanzione amministrativa. Cosa volete che siano, per una società di serie A che lotta per non retrocedere o per andare in Europa, 30.000 o La penalizzazione nella classifica, i punti tolti quando una società non fa quello che deve fare, le partite a porte chiuse lontani da casa; toccare gli interessi economici del calcio è l'unica sanzione che può riportare il calcio con i piedi per terra

Questo è lo sforzo che bisognerà compiere e, con la stessa lealtà e correttezza con cui votiamo questo decreto-legge, ci dichiariamo disponibili a proseguire per vedere cosa si possa fare insieme per il risanamento del calcio italiano, attraverso regole di fondo, a condizione che questo avvenga al di fuori di logiche di parte e nell'interesse della tranquillità del nostro sport ma, soprattutto, nell'interesse della società che viene falcidiata da atti di violenza intollerabili. Con questa impostazione e con il riconoscimento della continuità di questo provvedimento con quelli adottati dal precedente Governo Berlusconi e dal Ministro dell'interno di quello stesso Forza Italia esprimerà il proprio assenso alla conversione del decreto-legge al nostro esame. Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori e signori del Governo, il Gruppo dell'Ulivo, a nome del quale intervengo, esprime convintamente il proprio sostegno a favore del decreto-legge in esame sulla violenza negli stadi e attorno agli stadi. La situazione attuale è sotto gli occhi di tutti, non occorre in questa sede ripetere analisi e approfondimenti sulle cause di questa violenza. Quello che era uno splendido spettacolo si è trasformato in un problema di ordine pubblico, in un problema di sicurezza. Ed allora ben venga questo nuovo provvedimento del Governo che si pone l'obiettivo di porre un limite, dei freni alla violenza. Forse non è un caso che questa violenza si verifichi per lo più nell'ambito del mondo del calcio attorno e dentro al quale si scaricano tensioni sociali, economiche e politiche che hanno altra origine. Questo nuovo decreto-legge s'inserisce nella logica che già fu propria del decreto Pisanu, sicuramente positiva anche perché accolta e sostenuta - pure quella volta - dalla gran parte delle forze politiche. Il problema maggiore dopo l'approvazione di quel decreto è consistito nella mancata applicazione, almeno parziale, di una serie di norme di quel decreto stesso, particolarmente quelle relative alla sicurezza negli stadi e ai rapporti non sempre cristallini - per usare un eufemismo - tra alcune società e alcuni gruppi di tifosi. Proprio questo è uno degli obiettivi principali del nuovo decreto-legge: rendere concrete e applicare tutte le norme del decreto Pisanu, completare gli interventi nell'ottica della sicurezza, secondo le segnalazioni che ci sono pervenute dalle realtà e dai gruppi sociali che attorno al mondo del calcio vivono. Colgo l'occasione per dare atto dell'importante lavoro svolto dalle Commissioni congiunte giustizia e affari costituzionali e dai due colleghi relatori che, al termine di una serie di ampie e approfondite audizioni, hanno sintetizzo egregiamente le emergenze emerse. È stato molto positivo il lavoro svolto unitariamente dalle Commissioni congiunte, soprattutto per l'esame degli aspetti sia di natura repressiva che di formazione culturale dei giovani nell'ambito dello sport*,* come pure molto positivo è stato lo spirito con cui tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, hanno affrontato e risolto i punti nodali, i punti più delicati dell'intera vicenda. Va dato atto che in momenti e in situazioni di tensione sociale anche notevole, di emergenza, soltanto la collaborazione sincera e convinta di tutte le forze politiche può individuare e adottare le misura più adeguate alla soluzione dei problemi, di qualsiasi genere essi siano. Sicuramente rimangono degli aspetti irrisolti, come quelli relativi alla proprietà e alla gestione privata degli stadi, alla creazione di una sicurezza privata all'interno degli stadi, degli stadi, infine, alla responsabilità e alla previsione di sanzioni più efficaci nei confronti delle società sportive che non siano soltanto di natura pecuniaria, peraltro per importi che non fanno di certo paura alle grandi società. Ciò nondimeno, riteniamo e siamo convinti che le norme in via di approvazione in questa sede siano fondamentali nel tentativo di riportare il mondo del calcio nel giusto e corretto ambito in cui la violenza venga se non eliminata almeno ridotta e controllata il più possibile. In conclusione, riteniamo che la collaborazione piena e convinta di tutte le forze politiche per migliorare le norme originarie di questo decreto‑legge e l'attenzione che il Governo dovrà porre per l'applicazione di tutte le norme in materia possano costituire la migliore garanzia per l'ottenimento dei risultati che il decreto‑legge si propone.

***Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte***

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge costituzionale n. 1084, il cui testo risulta dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale presentati alla Camera nn. 193, 523, 1175 e 1231, è stato approvato all'unanimità dalla Commissione affari costituzionali del Senato e praticamente riguarda la modifica dell'articolo 27 della Costituzione in materia di pena di morte e allinea la normativa costituzionale alla normativa ordinaria prevista dalla legge 13 ottobre 1994, n. 589, che aveva espunto dal codice militare di guerra il richiamo alla possibilità di ricorrere alla pena di morte. La costituzionalizzazione del principio di abolizione rende impossibile per il futuro di potere reintrodurre la pena di morte sotto qualsiasi forma nel nostro ordinamento giuridico. Questo è il significato pratico, il significato concreto di questo provvedimento. Il disegno di legge in parola avrà bisogno come è facile comprendere, essendo un disegno di legge di modifica della Costituzione, ancora di due passaggi parlamentari, alla Camera dei deputati e al Senato.

L'approvazione di questo provvedimento legislativo, che è di rango costituzionale, è anticipata da molte sentenze della Corte costituzionale e anche da molte prese di posizione a livello politico e a livello sociale. Il provvedimento realizza il principio di tutela del bene fondamentale della vita che costituisce il più significativo dei diritti inviolabili dell'uomo, contenuto nell'articolo 2 della nostra Costituzione.

del 1930, sia pure per i delitti contro la personalità dello Stato e per i più gravi delitti comuni come la strage e l'omicidio aggravato. Fu soppressa dal codice penale dal decreto legislativo n. 244 del 1944 ed abolita definitivamente dall'articolo 27 della nostra Costituzione che, tuttavia, mantenne e mantiene ancora in vita (perché dobbiamo ancora approvare questo provvedimento

si afferma che la pena di morte non potrà essere più inclusa nel corpo delle leggi penali ordinarie e si conferma la tradizione giuridica italiana contro la pena di morte, ritornando alle luminose tradizioni italiane che ebbero in Cesare Beccaria l'apostolo e il maestro dell'abolizione della pena di morte.

una giuria infallibile». È inutile ricordare che questo provvedimento rende più credibile la richiesta del nostro Paese di ottenere una moratoria delle pene capitali nel mondo e rafforza il Trattato di Amsterdam del 1998, cui fu allegata una dichiarazione relativa alla pena di morte confermando l'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dell'inizio del 2000: tale articolo 2, al comma 2, con una norma di principio purtroppo non precettiva, ha stabilito che «nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato».

l'abolizione piena e senza condizioni della pena di morte, con una scelta che onora il nostro Paese e onora anche la tradizione di civiltà del popolo italiano.

visto che in Italia non si commina la pena di morte dal 1947. Ma definire nella Carta costituzionale il divieto di comminare questa sanzione per qualunque tipo di reato, anche militare, non è solo un atto simbolico. Non lo è in ragione del tempo in cui viviamo, che è, contro la nostra volontà, un tempo di guerra. Un tempo in cui, dopo la Guerra fredda, da un lato il crescere di un odioso terrorismo integralista e, dall'altro, la miope risposta della guerra permanente e preventiva ci disegnano uno scenario di conflitto, in cui quella parola odiosa, espunta dal vocabolario politico per decenni, torna ad essere pronunciata. Forse è destino che la memoria non si possa trasmettere con sufficiente forza, per cui, periti gli uomini e le donne che vissero con i loro occhi l'orrore delle bombe e le privazioni delle ostilità, oggi vengano meno la consapevolezza e il timore che ciascuno di noi dovrebbe avere nel pronunciare la parola «guerra». Ed è in questo scenario, in questo mondo, che affermiamo con convinzione che non è diritto di nessuno togliere la vita ad un altro uomo, né in tempo di pace né in tempo di guerra. Che affermiamo che anche nel legittimo uso della forza da parte dello Stato c'è un limite, il limite della vita. Quanta strada, quanti anni abbiamo dovuto aspettare dall'Assemblea costituente perché fosse matura la consapevolezza della necessità e dell'urgenza di questo passaggio. Quelle poche parole che oggi intendiamo togliere dalla Carta costituzionale ci riportano alla mente il conflitto della Prima guerra mondiale, la rotta dei nostri soldati, le parole di Cadorna riferite ai disertori: «Faccia fucilare, se occorre, immediatamente e senza alcun provvedimento, i colpevoli». Furono, secondo la Commissione d'inchiesta su Caporetto, 1.006 le condanne a morte. Ma chi erano quei morti dimenticati della Grande guerra? Erano contadini ed operai, buttati in una guerra che non gli apparteneva né capivano. E se oggi guardiamo a chi sono i condannati nei 54 Paesi che ancora praticano la pena di morte nel mondo, come allora, vediamo che sono la parte più debole del mondo, gli ultimi, gli emarginati, quelli che non hanno possibilità di riscatto. Non si tratta di alimentare un'insana e pelosa solidarietà per chi si è macchiato di gravi colpe, ma di riconoscere fino in fondo le conseguenze dell'ingiustizia sociale. Si pensi al caso più eclatante e visibile, gli Stati Uniti, la più grande democrazia liberale del mondo, quelli che si ergono a tutori del nuovo ordine mondiale. La Cina, certo, si macchia di orrendi crimini contro l'umanità, quando nel solo 2005 uccide più di 5.000 condannati a morte, così come l'Iran, secondo in questa classifica orribile. Ma certo il primo e più autorevole Paese occidentale è lo specchio delle contraddizioni della nostra cultura, e che il nostro modello fondato sul mercato porta con sé. Quel Paese, gli Stati Uniti, come l'Europa, assume il principio normativo della cecità di fronte al colore della pelle. Come l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea vieta la discriminazione razziale, così svariate sentenze della Corte Suprema affermano questo principio (e lo facevano già al tempo della segregazione razziale). Ma è davvero così? Negli Stati Uniti sono detenute 2.130.000 persone: si tratta di un record mondiale. Molti detenuti sono membri di minoranze razziali. Più precisamente: il 49 per cento della popolazione penitenziaria è composto da afroamericani, benché i neri siano il 12-13 per cento della popolazione. E se andiamo a verificare questi dati nella pena di morte, la selezione razziale è ancora più netta: uno studio del Dipartimento della giustizia ha mostrato che, dal 1995 al 2000, sono stati approvati 159 procedimenti per reati puniti con la pena di morte; il 72 di questi riguardava imputati appartenenti a minoranze razziali. Questi numeri, relativi al colore della pelle, sono ancora più chiari se andiamo a guardare l'appartenenza sociale di chi delinque. Credo che Credo che quella di oggi, signor Presidente e colleghi, sia una pagina importante e impegnativa per il nostro Parlamento, non un momento tra i tanti della vita dell'istituzione deputata a costruire le norme della convivenza civile. E proprio questo momento ci impone di assumere una consapevolezza che spero sia unanime. Le nostre istituzioni devono essere rigorose nell'applicazione della legge e nell'assicurare i diritti fondamentali dei cittadini, anche il diritto alla sicurezza. Ma non ci può sfuggire come la scelta di delinquere non sia, se non marginalmente, un fatto endemico dell'umanità, un accidente inguaribile: la gran parte dei delitti, anche quelli più truci e violenti, nasconde una domanda di benessere inevasa. Per questo, affrontare solo l'aspetto repressivo e non quello sociale della questione criminale è un approccio limitato e perdente. Chi delinque, paghi il dazio che la legge prevede, senza scorciatoie, ma lo Stato ponga le basi per ridurre quella drammatica emarginazione che porta a ritenere normale la scelta di delinquere. Lo dico pensando soprattutto alla condizione di vita dei migranti che vivono nel nostro Paese. un terzo dei detenuti è costituito da migranti. E questo non avviene certo - come vorrebbe qualche lombrosiano dell'ultima ora - per una naturale tendenza a delinquere, ma semplicemente perché, essendo esclusi dalle reti di protezione sociale, costoro vedono nel crimine l'unica possibilità di riscatto. Certo, non sempre i delitti sono motivati dal bisogno. Alcuni dei crimini più efferati che hanno scosso il nostro Paese in questi anni nascono con altre, spesso incomprensibili motivazioni. Cogne, Novi Ligure, Erba; basta citare i luoghi, neppure i nomi, per ricordare a noi tutti quegli efferati delitti. In tutte quelle occasioni abbiamo sentito commentatori e cittadini che dicevano: «Io sono contro la pena di morte, però...». Oggi diamo l'unica risposta che un Paese civile può dare: non c'è nessun «però». La civiltà di un Paese non si misura nei momenti più alti, ma di fronte alle tragedie più grandi, quando si è messi di fronte all'orrore, che pure esiste. La risposta è che c'è un limite alla punizione, la vita, e c'è una speranza di futuro anche per l'assassinio. E questo principio, che noi oggi certifichiamo con questo atto parlamentare, dev'essere un viatico importante perché divenga patrimonio condiviso dell'umanità tutta. Io voglio dare atto al Governo del suo impegno, prima confuso, ma presente, poi sempre più deciso, perché questo grande tema sia al centro dell'agenda politica mondiale. Le parole del presidente Prodi in quest'Aula, all'atto di chiedere la fiducia pochi giorni fa, sono un impegno che ci fa essere orgogliosi di appartenere all'attuale maggioranza. E la decisione di ieri del Consiglio d'Europa, grazie ad una caparbia volontà dell'Italia di dar vita ad una *task force* che agevoli le adesioni alla nostra proposta di moratoria, è un passaggio importante che spero verrà apprezzato in modo condiviso dall'intero arco costituzionale. Come già, in tanti, in quest'Aula abbiamo affermato in occasione della costituzione della Commissione parlamentare sui diritti umani, si apre di fronte a noi un percorso impegnativo, ma necessario: di fronte a chi ritiene possibile esportare la democrazia con la forza noi dobbiamo testardamente confermare l'affermazione dei diritti umani con l'energia della politica. In questo senso oggi può essere una bella giornata per il nostro Parlamento.

la senatrice Pellegatta ha già detto tutto, quindi rubo solo due minuti, ma ci tenevo moltissimo ad intervenire per portare, da quest'Aula, la piena solidarietà a tutti i disertori di tutte le guerre; volevo chiedere perdono per quelli che sono stati ammazzati da strutture di morte, da uniformi senza umanità e volevo portare un riconoscimento forte a loro e ai loro discendenti affinché questo non succeda più.

è la voce del loro nemico. E chi parla del nemico è lui stesso il nemico». Questa è una bella pagina per il nostro Senato, che accompagna anche l'iniziativa sulla fine della pena di morte

Signor Presidente, onorevoli senatori e senatrici, rappresentanti del Governo, il mio intervento non ha la pretesa, in questa discussione generale, di rappresentare l'opinione di un Gruppo parlamentare, è un mio contributo personale alla riflessione su un argomento sicuramente importante

che riguarda la condizione militare e la pena di morte, ed io voglio parlare più del principio che della tecnicalità della norma; e lo voglio fare sperando che oggi il Senato abbia la possibilità di riflettere seriamente seriamente sulla forza dei simboli, sulla forza anche della nostra storia come sistema Paese. Lo dico perché coincidenza temporale vuole che la Camera abbia trasmesso al Senato questo provvedimento l'11 ottobre 2006, cioè ben prima di fatti che hanno sconvolto l'umanità: mi riferisco a dittatori sanguinari che sono stati giustiziati; mi riferisco a Saddam Hussein; mi riferisco, cioè, all'utilizzo della pena capitale come strumento per fare giustizia. Il tema che introduce questo disegno di legge costituzionale è lo stesso che deve portare le persone, le comunità civili a rifiutare lo strumento della pena capitale come strumento per fare giustizia, e questo deve valere, evidentemente, non solo per le vicende e le questioni legate alla guerra, quelle legate alla fine di una dittatura, ma deve valere anche nella vita di relazione civile nel mondo. Signor Presidente, perché ho fatto riferimento a Saddam? Tutti noi ricordiamo che fu un triste Natale, l'opinione pubblica fu scossa, vedemmo immagini tremende in televisione; successivamente, ci fu chi ebbe più fegato e andò addirittura a curiosare sui siti Internet, per capire com'era avvenuto. Tutto questo provocò una repulsione nell'opinione pubblica mondiale; ci fu anche chi giustificò, sostenendo che è legittimo tutto (la mia posizione è esattamente opposta); ma credo che noi dobbiamo pretendere, sessant'anni dopo,

La barbarie c'è stata anche in questo Paese e a me ha fatto molto piacere leggere, qualche mese fa, una frase del ministro D'Alema che diceva quello che diceva a proposito di piazzale Loreto: anche quello fu un atto di barbarie. Non lo dico per nostalgia, lo dico per senso di civiltà, perché chiunque ha diritto ad essere giudicato, nessuno ha il dovere di giustiziare. Io credo che questo sia un fondamento che vorrei salisse dal Parlamento della Repubblica, proprio per gettarci alle spalle l'orrore della pena capitale in campo civile e in campo militare. Credo che questa sia una grande questione sulla quale l'Italia possa fare la sua parte. C'è un'altra questione collegata a questa, una questione di valori, c'è il grande tema della sacralità della vita che non può essere nella disponibilità di alcun giudice. Ecco perché sostengo convintamente la necessità di dare questo segnale, sia pure limitato ad una condizione di guerra, che può porre un altro tipo di problemi: pensiamo a quello che poteva accadere, durante i conflitti,

nemmeno quello che succede ancora oggi, non più in Italia, non più per responsabilità dell'Italia in riferimento ad atti sottoposti al codice di guerra in tempo di pace,

costituzionale, su come mobilitare l'opinione pubblica mondiale - non bastano le comparsate alle Nazioni Unite alla ricerca di voti, occorre una politica che possa condizionare effettivamente l'abrogazione di questo strumento incivile

Questa è una questione che esiste e vorrei che il Parlamento rispondesse. Faccio un esempio: quanto deve prevalere ancora un senso dell'economia sull'affermazione di un dovere di civiltà? Quanti sono i Paesi con i quali intessiamo relazioni economiche che praticano la pena di morte? C'entra o no, in questa discussione, anche il dibattito sul tema delle prospettive delle economie nel mondo? Vorrei sapere se c'è un dato certo sui Paesi che praticano la pena di morte e vorrei sapere con quanti di questi Paesi abbiamo rapporti economici, ad Est come ad Ovest. Lo ripeto: ciò riguarda le democrazie e le teocrazie, non riguarda una categoria di particolari Stati nazionali o federali. Quando - per citare una frase cara a Papa Wojtyla - l'universalizzazione delle garanzie avrà finalmente la prevalenza sulla globalizzazione dell'economia? Anche questa questione credo ci debba far interrogare: è un tema grande, signor Presidente. Credo che il legislatore ordinario e il Governo debbano fare la loro parte per non consentire mai più che la pena capitale sia strumento per praticare giustizia.

membri del Governo, oggi votiamo un bel provvedimento con una maggioranza coesa, finalmente, in cui avremo finalmente un premio della bontà: abbiamo cancellato la pena di morte in caso di guerra, e andrà su tutte le pagine dei giornali della sinistra come la vittoria della pace.

caso di guerra è presente in Afghanistan. L'uso della forza è in qualche modo consentito per la difesa o possiamo opporre semplicemente un atto di buona volontà?

uccidono regolarmente tutte le donne colte o, quantomeno, che sappiano leggere e scrivere e stuprano gli altri. Ebbene, con queste persone voi volete fare il tavolo per la pace: per la pace: a queste persone dobbiamo mandare l'esercito! Non si trattava con Hitler; non si tratta con i talebani. Ad Hitler e ai talebani si manda l'esercito. Oggi noi Oggi noi approveremo un primo passaggio costituzionale, allora io dico: viva l'ipocrisia! Qui la vita viene ben colta, ma ci sono - come ha detto anche il collega Storace - altri momenti in cui la vita per voi non ha la medesima sacralità, non proviene dal medesimo principio, cioè che la libertà e la vita non sono nelle disponibilità dello Stato. Stiamo discutendo in questi giorni, nel silenzio,

«Welby non ha nessuna possibilità di migliorare»; anche noi non abbiamo possibilità di migliorare, ahinoi, perché l'orologio biologico ci porta inevitabilmente verso la conclusione. Marino

«Exit», l'associazione per il diritto ad una morte dignitosa (perché la morte non si chiama più morte, ma pietà,

(su cui sicuramente la pietà e i buoni sentimenti del centro-sinistra si sprecano) comprendesse la possibilità di ricorrere all'eutanasia o al suicidio assistito. Infatti, dicono che oggi i medici intervengono per assistere alla fase terminale della vita attiva e passiva. Questa è vita o non è vita, signor Presidente? Oppure torniamo al concetto della vita degna di essere vissuta,

Parliamo poi di altri condannati a morte dall'ipocrisia. Questi sono condannati a morte dal vostro buonismo e dalla vostra pietà, di cui, vi prego, fatecene ammenda. Non abbiate più pietà dei malati. Lasciateli stare, lasciateli alle famiglie! Lasciateli ai medici. Risparmiate loro la vostra pietà!

Altra ipocrisia; altri condannati a morte dall'ipocrisia, e ne cito solamente uno:

persone che non avevano ancora finito di compiere il percorso di riabilitazione e di pagare il proprio debito con la giustizia,

Oggi questo provvedimento, che voi sbandiererete domani, incorniciato da varie bandiere della pace, è un atto di ipocrisia evidente.

condannato all'interruzione volontaria di gravidanza e che in tutti quei casi sussistano condizioni di urgenza per la salute psichica o fisica della donna o del nascituro. C'è qualcosa che non funziona. Questo numero di aborti è una sconfitta per tutti; prima di tutto per le donne. Ebbene, su questi temi di attaccamento alla vita vorremo vedere una discussione seria,

almeno direttamente (anche se lo siamo già in modo asimmetrico con una consistente parte dell'Islam), ma si preoccupi anche di questi altri condannati a morte per l'indulto, per l'aborto e anche anche per l'eutanasia, che è una pietra tombale da parte dei buonisti di questa maggioranza coesa, coesa, coesa. *(Applausi

delicata materia ha lasciato libertà di coscienza; pertanto, ognuno potrà fare dichiarazioni a nome proprio e voterà - ripeto - secondo la propria coscienza. Quello che ha fatto specie, Presidente, è che su questa materia siano intervenuti quattro disegni di legge temporalmente diluiti, ma che avevano lo stesso, identico testo. Questo ci ha fatto capire che non era opportuno ripresentare disegni di legge che non differivano neanche di una virgola dal precedente. A questo punto, vien da pensare che c'è stata una corsa ideologica c'eravamo, anche noi su questo tema abbiamo presentato la nostra proposta» che, guarda caso, era perfettamente identica alla precedente. Questo ci fa pensare che ci sia poca seria intenzione, se non quella di sbandierare ideologicamente un provvedimento che, dobbiamo ricordare ai colleghi di sinistra, è del tutto inutile del tutto inutile perché la pena di morte nell'ordinamento italiano non c'è, non esiste. Esiste soltanto un refuso nell'articolo 27 che non tiene conto del contesto del sistema per cui sembrerebbe che, in caso di guerra, il codice militare di guerra potrebbe reintrodurre la fatidica pena di morte.

che andava a risolvere! Non si è voluto inserire un requisito importantissimo fra le condizioni impeditive dell'applicazione dell'indulto: la verifica della pericolosità sociale di chi si andava a liberare; ci si è fermati esclusivamente ai limiti temporali della pena comminata. Guardate che nessun magistrato può procedere alle misure alternative prescindendo dalla valutazione della pericolosità sociale. Questo Parlamento ha liberato metà carceri italiane non considerando la pericolosità sociale. Il mio collega ha ricordato una delle poche decine di vittime che questo Governo ha sulla coscienza. La pena capitale è stata reintrodotta con quella nefasta norma che ha consentito l'indulto nel nostro ordinamento. Questa è la pura verità. Pertanto, per una questione di responsabilità, per una questione di non dare corpo a ciò che corpo non ha, perché è un pretesto e solo una pulizia legislativa - ripeto - che non modifica assolutamente nulla di sostanziale nell'ordinamento italiano, il sottoscritto, che purtroppo può solo parlare a nome personale, non voterà questo provvedimento, ma si asterrà.

in piena coscienza e non senza qualche imbarazzo, perché nella passata legislatura quantomeno in Commissione votai a favore, a favore, qualche perplessità perché troppo sbrigativamente si risolve l'oggetto del disegno di legge come se nel nostro ordinamento oggi vigesse la pena di morte o, meglio, come se nel nostro ordinamento costituzionale oggi fosse ammissibile la pena di morte. Questo l'articolo 27 della Costituzione

Il punto è che la nostra Costituzione prevede un'eccezione al divieto costituzionale dell'ammissibilità della pena di morte.

che non comporta l'obbligo per il nostro ordinamento di dotarsi di questa sanzione estrema, radicale, addirittura disumana, ma consente al legislatore

che la Nazione italiana sia in stato di guerra (stato che, come è noto, deve essere dichiarato con le guarentigie previste dalla Carta costituzionale).

eletto dai suoi cittadini in modo democratico, debba precludersi la possibilità, di fronte ad un'emergenza di guerra,

quanto meno in funzione di deterrenza. Ho ascoltato l'inno alla diserzione del collega Silvestri,

Presidente, responsabilmente e facendo appello alla mia coscienza, non so se unirò il mio voto a quello dei colleghi che, immagino, in stragrande maggioranza o quasi all'unanimità approveranno questo disegno di legge. In coscienza, devo pormi questo problema

determinare gravissime ripercussioni sull'incolumità di migliaia e migliaia di persone e sulla stessa conservazione dello Stato di diritto.

in cuor mio, di precludere a questo Parlamento di ricorrere - Dio non voglia - a una previsione del genere con le garanzie previste dalla nostra Costituzione.

perché sembra che vadano avanti le bandierine ideologiche, piuttosto che le questioni serie. Oggi abbiamo letto sul principale quotidiano italiano la notizia che, a seguito di un intervento abortivo, un bambino è nato vivo e vitale, anche se in pessime condizioni, come è ovvio. Il nostro ordinamento non tutela la vita umana innocente, tant'è che è possibile l'aborto a richiesta; non tutela la vita umana nelle sue fasi critiche, se è vero che l'autorità giudiziaria archivia un caso di patente eutanasia, dopo che una commissione, nominata dal Ministro della salute in carica, ha accertato che non vi era alcun accanimento terapeutico. Ci si attenderebbe una riflessione ampia su tutto questo, ma tutto questo non è seguito da riflessione ampia. Tante donne extracomunitarie, la maggior parte appartenenti a comunità di matrice islamica, presenti in Italia, subiscono vessazioni, violenze e talora anche la morte per atti che in qualunque Paese civile sarebbero normali e in questo momento, invece, la priorità sembra essere un'altra. Non vi è un tempo di guerra in atto, non vi è un tempo di guerra a breve - grazie a Dio! - e neanche a medio e lungo termine.

che non sono reali né attuali, ma che sono esclusivamente ideologiche. Soprattutto, non riesco a condividere, a fondamento di certe proposte, un inno alla diserzione nel momento in cui nostri uomini in divisa difendono la pace in tanti scenari internazionali. Per questo motivo non parteciperò al voto.

è una legge di senso, nel senso che finalmente, con pieno diritto, saremo un Paese abolizionista e con pieno diritto potremo portare all'interno dell'ONU e di tutte le altre sedi preposte la volontà del nostro Paese di essere contrario alla pene di morte, comunque e in ogni luogo. Questo è un passaggio importante proprio perché tutta la società prende una decisione che va in una direzione chiara rispetto al concetto di morte, soprattutto se legato ai fatti che riguardano la pena di morte militare. Ho condiviso, ad esempio, al contrario di altri, l'intervento

del nostro Paese su diversi fronti. E anche questo assume un significato ulteriore; è un'apertura rispetto anche ad altre civiltà che deve essere perseguita coerentemente arrivando fino alle estreme conseguenze da questo punto di vista, cioè mettendo in discussione anche quelli che sono comunque strumenti di morte, come le guerre e quant'altro. Credo che la società oggi debba trovare la forza ed il carattere per per riuscire ad affrontare con altre modalità le tensioni esistenti sull'intero pianeta. E come fare se non partiamo dal nostro territorio e, soprattutto, dalla pulizia non solo formale

*(UDC)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, quella di oggi è una data importante per il nostro Paese poiché viene abolito definitivamente qualsiasi riferimento alla pena di morte nel nostro ordinamento giuridico-costituzionale. La modifica dell'articolo 27 della nostra Carta costituzionale, con la soppressione del quarto comma, elimina infatti, in via definitiva, anche il riferimento ai casi previsti dalle leggi militari e di guerra. Con questa modifica anche l'Italia può chiedere con maggiore forza l'abolizione della pena di morte nei Paesi in cui è ancora vigente. L'UDC vota convintamente a favore del provvedimento in esame, un provvedimento di civiltà, a difesa della vita che va considerata importante sempre e comunque, dall'atto del concepimento fino alla morte naturale. La pena di morte rappresenta l'atto punitivo più estremo che non racchiude in sé nessuno degli elementi di recupero e rieducazione del soggetto che ha commesso reati anche gravi. Non è certo attraverso la pena di morte che si prevengono fenomeni di criminalità. Il Paese che ha dato i natali a Cesare Beccaria non poteva che approvare in via definitiva l'abolizione di questo riferimento alla pena di morte, come grande atto di civiltà che fa onore a tutto il Parlamento.

Signor Presidente, anche il mio Gruppo è pienamente favorevole all'abolizione della pena di morte, quanto meno a questo residuo di pena di morte iscritto nell'articolo 27 della Costituzione.

po' Bobbio, che, se ci dovessimo dilungare a pesare i pro e i contro della pena di morte, non finiremmo mai perché ci sarebbe sempre la prevalenza di qualche elemento sia pro che contro. Alla fine, però, bisogna dire che questo circolo vizioso di morte che innesca altre morti deve essere interrotto in una sua parte, e chi lo può interrompere è proprio quell'organismo che detiene una moralità superiore, cioè lo Stato. È lo Stato che per primo deve dire no alla pena di morte, che per primo deve dare l'esempio per affermare, appunto, che non si può punire con questa pena estrema. Credo che l'Italia non possa in questo momento non eliminare dalla Costituzione tale residuo, anche perché non può legittimamente chiedere ad altri Paesi l'abolizione della pena di morte mantenendone

a nome del mio Gruppo che, peraltro, ha lasciato sostanziale libertà di coscienza ai propri componenti. Vorrei però sottolineare, come hanno già fatto in maniera compiuta i colleghi Polledri e Divina, la sostanziale ipocrisia di quello che stiamo per fare oggi, nel senso che è ovvio che, in linea di principio, siamo tutti contrari alla pena di morte, anche nei casi più estremi, rispetto ai quali, peraltro, magari un minimo di attenzione la si dovrebbe comunque mantenere. Ricordo, però, che, anche se in Costituzione marginalmente è rimasta come residuo, in realtà, la legislazione corrente del nostro Paese ha già abbondantemente, da moltissimo tempo, superato la questione nel senso che, di fatto, dal punto di vista puramente legislativo, nel nostro Paese oggi è già impossibile procedere ad un'esecuzione capitale. Vorrei sottolineare però quanto non detto in quest'Aula, nel senso che, come si è fatto su moltissimi altri argomenti, ci ci si concentra e si porta avanti, con grande enfasi, l'azione parlamentare su situazioni ormai sostanzialmente di dettaglio e si fa finta di non vedere

limitarsi, nella sua azione, nella sua visuale, alle uniche cose che sul momento gli possono far comodo. Se vogliamo parlare di pena morte,

Quindi, a fronte di una pena di morte ufficiale che nel nostro Paese di fatto non esiste, non si può non parlare delle altre pene di morte che invece nel nostro Paese vengono

alla legge che regolamenta l'interruzione di gravidanza, rispetto alla quale, come ha già detto il mio collega Polledri, noi non siamo minimamente contrari ai principi istitutivi, però certo attuazione quotidiana ha qualcosa nei numeri che evidentemente non quadra. Qui però passano gli anni, passano i decenni ed è un argomento che, nel rispetto del politicamente corretto, si continua a non affrontare e questa è cosa non giusta. Ricordo la questione dell'indulto, che non ripeto. Ricordo anche la questione degli appartenenti a gruppi terroristici nel nostro Paese che hanno compiuto, loro sì, esecuzioni capitali di morte nei confronti di altri cittadini che oggi addirittura ospitiamo nelle nostre istituzioni. A questo proposito, sono perfettamente d'accordo che una volta che una persona ha espiato la colpa è di nuovo un libero cittadino, ma credo che una colpa come l'omicidio non si possa considerare espiata dopo otto, dieci, dodici anni, come invece sta avvenendo nel nostro Paese. Inoltre, se rispetto alla pena originariamente prevista, con l'assurdità che esiste nel nostro Paese, si ha una riduzione della metà, di un terzo, dell'80 per cento, non possiamo ritenere espiata la colpa, possiamo eventualmente ritenere anticipata l'uscita dal carcere ma, di fatto, dal punto di vista morale, quelle sono persone che la loro colpa ancora non l'hanno espiata.

però siccome poi c'è il tornaconto economico o semplicemente il politicamente corretto si fa finta di nulla. Abbiamo mandato migliaia di rappresentanti, dal Primo ministro in giù, in un paese come la Cina, che da sola fa il 90 per cento delle esecuzioni capitali

Esistono poi soprattutto decine e probabilmente centinaia di Paesi, che non hanno l'onore della cronaca semplicemente perché non sono seguìti dalla televisione, dove nell'oscurantismo più assoluto le esecuzioni capitali avvengono quotidianamente; non rientrano neanche nella statistica

Quindi, sarei stato portato ad esprimere un voto contrario proprio per l'ipocrisia che il provvedimento oggi in esame ha rappresentato in quest'Aula. Non mi esprimo in tal modo perché mi rendo conto che ciò potrebbe essere strumentalizzato e considerato una posizione favorevole alla pena di morte. Evidentemente, non è così; tuttavia, onestamente, al di là di un voto di astensione che è sostanzialmente un voto di protesta contro l'ipocrisia che anche stamani abbiamo verificato in quest'Aula, non posso andare.

L'articolo 27 della Costituzione già non ammetteva la pena di morte, salvo nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

quanto accaduto in Iraq alcuni mesi fa, dopo aver visto la scena alla televisione dell'impiccagione di Saddam

Affrontando questo tema abbiamo tutti la consapevolezza di affermare un principio di altissimo significato etico. Infatti, l'abolizione della pena di morte è argomento che da secoli interroga le coscienze della civiltà giuridica occidentale. La modifica costituzionale sottoposta oggi all'esame del Senato - per la quale anche chi parla aveva presentato una propria proposta di legge, sottoscritta da altri autorevoli esponenti di Forza Italia - prevede la cancellazione di ogni riferimento alla pena di morte nella Costituzione. Con tale iniziativa abbiamo inteso dimostrare che c'è un *idem sentire* anche nel Paese, che va al di là e supera gli steccati degli schieramenti politici predefiniti. Invero, su questo tema anche in passato le forze politiche hanno saputo trovare una proficua intesa di tutto il Parlamento. Voglio ricordare in proposito le iniziative assunte nelle scorse legislature che non sono giunte a buon fine e voglio ricordare in particolare il voto pressoché unanime della Camera dei deputati nel corso della XIV legislatura, in data 4 giugno 2002, che però non ha trovato seguito proprio presso questo ramo del Parlamento. Abbiamo la speranza, quindi, che la XV legislatura repubblicana possa portare alla definitiva approvazione di questa importante riforma costituzionale: è la concezione personalistica dell'uomo che ritiene inaccettabile la pena di morte e che affonda le proprie radici nell'Umanesimo, sia cristiano sia liberale. Voglio ricordare che il primo Stato ad abolire la pena di morte fu il Granducato di Toscana, con una legge risalente al 1786; dopo l'Unità d'Italia, la pena capitale fu soppressa nel codice penale del 1889 e ripristinata soltanto dal regime fascista nel codice penale del 1930; l'ultima esecuzione capitale nel nostro Paese ha avuto luogo a Torino, il 4 marzo 1947, e la pena di morte è stata, quindi, espunta dal nostro ordinamento dall'articolo 27 della Costituzione, che l'ha prevista soltanto nei casi previsti dalla leggi penali militari di guerra. Ricordo ancora, però, che, già nel corso del dibattito svolto all'Assemblea costituente, aveva trovato ingresso la tesi, all'epoca rimasta minoritaria, che propugnava la soppressione, nel nostro ordinamento, della pena di morte senza alcuna eccezione, anche nei codici militari. In tal senso ed a tal proposito, voglio ricordare in particolare la posizione assunta da Pietro Mancini. Anche il Concilio Vaticano II, nell'enciclica «*Gaudium et Spes*», a sua volta, ha condannato, come violazione dell'integrità della persona umana, le torture inflitte al corpo ed alla mente, rigettando senza riserve tutto quanto è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio. Peraltro, già nel 1994, a seguito dell'approvazione della legge 13 ottobre 1994, n. 589, la pena di morte è stata espunta dal codice penale militare di guerra sul piano giuridico, un particolare significato è da attribuire all'ormai storica sentenza n. 293 del 1996 della Corte costituzionale. Questa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme attuative dei trattati di estradizione con la Francia e con gli Stati Uniti, nella parte in cui consentivano l'estradizione di persone incriminate per delitti puniti in quei Paesi con la pena capitale, anche in presenza di assicurazioni e impegni a non dare esecuzione a pene capitali. Le conseguenze di tale pronuncia sul piano giuridico sono addirittura paradossali: di fatto, oggi, l'estradando gode di garanzie più ampie, circa la non applicabilità del supremo supplizio, rispetto a quelle godute dal cittadino italiano che venga a trovarsi in uno stato di guerra, il che riteniamo sia un assurdo. È per questo motivo che ritengo che l'iniziativa parlamentare in esame, di profondo valore e significato, vada ad accompagnarsi all'azione che il nostro Paese ha intrapreso in ambito ONU per una moratoria delle esecuzioni delle pene capitali nel resto del mondo. Contrariamente a quanto è stato anche sostenuto nel presente dibattito, la proposta oggi in esame non è soltanto una petizione di principio. In un futuro, infatti, nessuna legge ordinaria potrà più ripristinare la pena di morte: se tale modifica non venisse attuata, in caso di eventi bellici, sarebbe assai agevole modificare la legge n. 589 del 1994 e sarebbe sufficiente, magari, solo un decreto-legge per ripristinare la pena capitale; viceversa, la sensibilità sociale e religiosa del nostro Paese, ormai, considera tale sanzione come contraria ad un dettato etico che non può trovare in nessuno caso deroghe: nessuno può privare un altro uomo della vita, bene supremo tutelato dall'articolo 2 della Costituzione. È del tutto evidente, inoltre, l'intimo contrasto esistente nell'attuale disposto dell'articolo 27 della Costituzione: in effetti, come può tendere alla rieducazione del condannato una pena che lo priva addirittura del bene supremo della vita? Come potremmo mai affermare che la pena capitale è un trattamento conforme al senso di umanità? Va, peraltro, considerato che il nostro Paese ha sottoscritto trattati internazionali che pure lo invitano ad abolire del tutto la pena di morte. Questa, dunque, viola il diritto alla vita; è stato provato che non ottiene alcun effetto dissuasorio rispetto alla commissione di reati ed è foriera di ingiustizie gravissime (è il caso di errori giudiziari, purtroppo irreversibili, soprattutto in tempo di guerra). Al di là, però, di queste ultime motivazioni di ordine pratico e giuridico, ci spingono a sostenere convintamente la proposta di legge al nostro esame ragioni di ordine morale ed etico. Quindi, o che si faccia riferimento ad un credo religioso o, più semplicemente, ad una fede laica, riteniamo doveroso affermare i principi della centralità e della dignità dell'uomo, unico ed irripetibile, e dell'intangibilità della vita umana. A nostro giudizio, lo Stato non può essere giustiziere e, nel contempo, deve porsi l'obiettivo di esercitare una giustizia mite, equa e non vendicativa: è con riferimento a questi alti principi di natura morale, storici, giuridici, fatti di misura e limiti e che appartengono alla tradizione culturale del nostro popolo, che Forza Italia sostiene convintamente la proposta di cancellazione della pena di morte dalla Carta costituzionale del nostro Paese e che, quindi, esprimerà voto favorevole. *(Applausi

signor Presidente, quel corpo di norme che la sinistra ha sempre ritenuto immodificabili anche rispetto alle recenti vicende sulla revisione costituzionale e che oggi invece viene toccato con questa modifica. Va ricordato che proprio l'ultimo comma dell'articolo 27 fu approvato dai Costituenti senza alcuna modifica e senza alcuna osservazione, a dimostrazione che su quel comma non ci fu travaglio tra le grandi forze che elaborarono il progetto costituzionale, che riguarda diritti e doveri dei cittadini e nel titolo fa appunto riferimento ai rapporti civili. Signor Presidente, sono contrario sempre alla pena di morte, sono altresì contrario, però, al metodo che è stato seguito, sono contrario all'eutanasia, sono contrario all'aborto, sono favorevole alla vita fin dal concepimento, ma su questo la sinistra ha certamente posizioni diverse. Non si può essere favorevoli alla vita a giorni alterni. Non abbiamo visto cortei della sinistra sulla pena di morte applicata in Cina o in tanti Paesi islamici, e in tanta altra parte del mondo dove le esecuzioni sono all'ordine del giorno. signor Presidente, di quella ragazza pakistana che viveva a Brescia non era una condanna a morte? Non abbiamo visto né cortei, né indignazione. Per queste ragioni,

per la pena di morte che ha espresso, a nome di Alleanza Nazionale, il mio Capogruppo, il senatore Matteoli, in questo caso non mi sento di confondere il mio voto con chi, in quest'Aula, ha fatto l'apologia dei disertori e soprattutto non mi sento di privare, per principio, la Nazione italiana di uno strumento

Signor Presidente, in Italia per la prima volta la pena di morte fu abolita nel 1889 con la promulgazione del codice Zanardelli. Fu reintrodotta nella tragica fase del regime fascista, per poi essere nuovamente cancellata il 27 dicembre 1947, con la promulgazione della Costituzione repubblicana.

Il 13 ottobre 1994 è stata promulgata la legge n. 589, che ha cancellato la pena di morte dal codice penale militare di guerra, l'Italia è così diventata un Paese totalmente abolizionista. In questo contesto di convinto contrasto nei confronti della pena di morte, si pone la proposta di modifica costituzionale che stiamo discutendo e che è stata così attentamente presentata dal collega Saporito. L'approvazione della modifica dell'articolo 27 della Costituzione è il punto d'arrivo di un comune percorso culturale e politico che appare doveroso per i parlamentari di un Paese democratico fondato sui diritti dell'uomo. La coscienza dell'inviolabilità dei diritti umani è comune alle forze politiche presenti in Parlamento e fa parte del patrimonio dei valori della grande maggioranza dei cittadini italiani. Il principio di tutela assoluta del diritto alla vita è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo tutelati dall'articolo 2 della Costituzione. Successivamente, il nostro Paese ha ratificato la Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre del 2000, che prevede all'articolo 2 che: «Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato», e all'articolo 19 19 che: «Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti». Credo che Credo che proprio per questo dobbiamo precisare ai colleghi intervenuti, al collega Silvestri da un lato, ai colleghi Pastore e Mantovano dall'altro, che qui non si tratta di discutere della diserzione, che resta un reato nel nostro ordinamento. Il nostro ordinamento, tra l'altro,

dai rischi paventati. Contemporaneamente, vorrei rassicurare i colleghi Polledri e Divina che né l'eutanasia, né il suicidio assistito sono mai stati oggetto dell'azione o dell'iniziativa del Gruppo dell'Ulivo e del centro-sinistra, come testimoniano ampiamente i lavori della Commissione igiene e sanità e come sempre è stato escluso in questo Parlamento. Il problema che abbiamo da affrontare e risolvere oggi, dal punto di vista giuridico, è estremamente semplice: il testo vigente dell'articolo 27 della Costituzione recita al quarto comma: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». Dalla volontà di risolvere questo problema nasce il testo approvato dalla Camera dei deputati, che ha l'obiettivo di cancellare dalla Costituzione anche il riferimento alla pena di morte come eventualità che può essere prevista dalle leggi militari di guerra. Eravamo ad un passo dall'approvazione di questa importante modifica costituzionale già nella passata legislatura e un altro tentativo si fece nella XIII. Oggi, siamo qui per compiere l'ultimo atto formale di un'azione positiva e lunga del nostro Paese nella direzione della completa cancellazione della pena capitale dal nostro ordinamento. Con l'approvazione di questo atto saremo più forti e più autorevoli nel sostenere, nei confronti degli altri Paesi, l'abolizione della pena di morte e la moratoria universale nei confronti delle esecuzioni capitali, che abbiamo avanzato presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il presente disegno di legge è in assoluta continuità con l'azione svolta dal nostro Paese, dal Parlamento italiano e in particolare dal Senato, il quale, nelle passate legislature,

si è battuto per l'abolizione della pena di morte e per una moratoria delle esecuzioni capitali, approvando in Parlamento, in più occasioni, chiare ed impegnative risoluzioni e rivolgendosi ad altri Paesi per allargare il campo delle Nazioni che sceglievano, di diritto e di fatto, l'abolizione della pena di morte. Ecco perché,

sullo stesso argomento è intervenuto l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Moretti, che ha dato tutte le garanzie possibili ai rappresentati della Regione Umbria. Una cosa bella - per carità - e positiva, però, mi sembra strano che il Governo,

su quanto apparso sulla stampa siciliana ieri: una forte preoccupazione circa il disegno di Trenitalia di abolire il traghettamento dei treni

se i treni non dovessero più essere imbarcati sui traghetti. L'ipotesi è di far risparmiare alle Ferrovie dello Stato 150 milioni di euro e poi trasportare i passeggeri con i bagagli da Villa San Giovanni a Messina e viceversa con aliscafi. Riteniamo che la Sicilia non possa assolutamente subire tale penalizzazione. Pertanto, prego

finestra"). Questo sarà senz'altro fatto. Mi permetto soltanto di suggerirle di assumere l'iniziativa di uno strumento ispettivo formale, in modo tale da sollecitare la

per una grottesca accusa di calunnia. Ho appreso oggi che le persone che egli ha consentito

mentre lui, che ne ha consentito l'arresto grazie alle sue puntuali segnalazioni, si trova in carcere per calunnia nei confronti non di queste persone - perché evidentemente erano davvero

per essere arrestato, chiedendo che venissero accertate bene le fonti di quanto egli avrebbe detto. Credo che un Ministro della giustizia non dovrebbe entrare nel merito di una vicenda giudiziaria riguardante una persona, ma dovrebbe invece rispondere alle interrogazioni e controllare

che sarebbe stata disposta dal ministro Amato, per sua stessa dichiarazione, nei confronti della Commissione parlamentare, a sua volta di inchiesta, sul

di dominio pubblico che è all'attenzione della Giunta per le elezioni. Direi che una serie di violazioni così gravi e di dichiarazioni inquietanti da parte del ministro Mastella e del ministro Amato meriterebbero,

Senatore Malan, anche per quanto riguarda le sue sollecitazioni, l'impegno della Presidenza è di darvi seguito e quindi di far giungere a conoscenza della sua

Signor Presidente, vorrei chiedere ancora una volta che il Ministro dell'interno venga a rispondere a una serie di interrogazioni che riguardano la sicurezza della città di Roma. Il Ministro si interessa molto della sicurezza in ogni parte d'Italia, ma, vivendo egli a Roma, dimentica che c'è un problema di sicurezza anche nella nostra città. Un mese e mezzo fa, sono sono stati aboliti i pattugliamenti notturni della Polizia di Stato per mancanza di mezzi, proprio in zone dove poi si sono verificati atti gravi di banditismo, come assalti a supermercati e attività commerciali.

per vedere che cosa stava avvenendo. Credo che il Ministro dell'interno debba rispondere di queste situazioni, anche perché i consiglieri comunali sono stati eletti dai cittadini e meritano tutta l'attenzione e il rispetto da parte delle forze dell'ordine.

che è uno strumento fondamentale della politica economica soprattutto nel settore della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e che rappresenta 120 miliardi di euro della spesa complessiva del bilancio delle pubbliche amministrazioni. Il piano di riassetto e ristrutturazione organica della società pare sia stato approvato solo a maggioranza con parere contrario del collegio sindacale. Vorremmo pertanto sapere dal Ministro dell'economia se condivide questa linea strategica o se, almeno, sia a conoscenza

che, a larghissima maggioranza, hanno deciso di trasferirsi dalla Regione Marche per essere aggregati alla Regione Emilia-Romagna. Il *quorum* raggiunto è stato notevole, pari al 67 per cento, con una percentuale di sì corrispondente all'83,91 per cento dei votanti. Il risultato é stato pubblicato regolarmente sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre del 2006. In funzione del combinato disposto dell'articolo 45, della legge del 25 marzo 1970, n. 352, e dell'articolo 132, della Costituzione, il Ministro dell'interno, entro i successivi 60 giorni, avrebbe dovuto presentare un disegno di legge ordinaria. 28 dicembre al 26 febbraio; il Ministro dell'interno non ha rispettato questo termine che peraltro, come si sa, è ordinatorio e non perentorio. perentorio. Mi permetto di sollecitare il Ministro per conoscere non soltanto le ragioni di questo difficilmente spiegabile ritardo, ma soprattutto quando presenterà in Parlamento il disegno di legge previsto dalla legge ordinaria che fa riferimento alla Carta costituzionale. sicuramente in modo di sollecitare il Ministro dell'interno rispetto all'interrogazione da lei presentata e praticamente illustrata.